Signor Presidente, desidero sollevare una questione che sottopongo alla sua attenzione affinché ne possa parlare nel Consiglio di Presidenza, nella Conferenza dei Capigruppo e per qualche riflesso anche nella Giunta per il Regolamento.

non solo complicato, ma addirittura impossibile sapere quale sia il testo finale che il relatore ha in mente, ovvero il filo conduttore lungo il quale si svolgerà non solo la discussione generale, ma anche l'opera emendativa da parte del Senato. Presidente, ciò è - lo ripeto - rispettoso del Regolamento e della prassi, però non funziona, perché un collega che voglia leggere il testo finale in maniera armonica e semplice praticamente non lo può fare. che cosa si possa fare: mi affido alla bravura, alla solerzia, alla qualità della nostra burocrazia interna che sicuramente saprà trovare una soluzione.

in maniera informale si può chiedere ai relatori di allegare alla loro relazione il testo che secondo loro dovrebbe essere approvato; così non si modificherebbe né la prassi né il sia utile trovare un modo per dare ai colleghi la possibilità di leggere senza troppe complicazioni il testo che almeno il relatore (non dico la Commissione o l'Assemblea, perché questo lo sapremo solo quando andremo a votare) ha in mente,

signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, se mi permettete, prima di entrare nel merito del provvedimento anch'io vorrei tentare di dare una risposta al collega Boccia che ha posto una questione sulla quale tutti ci siamo interrogati.

intestati al lavoro collettivo e non già ai singoli presentatori. Questa è l'unica traccia che abbiamo e che ci dà il segno visibile del lavoro da noi compiuto. Non c'è più l'identificazione dei presentatori

Il Governo ha dato una risposta tempestiva, ritenendo appunto di dover fornire un quadro di norme certo, un quadro di norme nuovo, non in contrasto con le misure precedenti ma in piena coerenza con il decreto Pisanu del 2003, cercando ovviamente di adottare tutti quei miglioramenti, quelle misure

agli avvenimenti sportivi e alla presenza assai fastidiosa di gruppi di persone molto spesso legate ad associazioni anche di tipo criminale. Riguarda anche la possibilità di controllare più segnatamente l'identità

personale introdotto con riferimento all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quanto ai requisiti, ricordo che nei decreti attuativi del decreto Pisanu del 2003

Il comma successivo riguarda la mera detenzione di questi arnesi. L'articolo 4, procedo assai rapidamente, riguarda le possibilità di arresto.

I due elementi sui quali verteva all'epoca la questione erano se l'arresto poteva essere differito e quali elementi potessero essere utilizzati. All'epoca, noi sostenevamo che l'arresto differito non era una problema ma che poteva esserlo l'utilizzazione di prove diverse da quelle fotografiche e audiovisive. Qui, in buona sostanza, viene recuperata quell'antica ispirazione dell'opposizione, non me ne vogliano i colleghi dell'opposizione attuale, alla quale si eliminano le prove successive ma si amplia il termine ai fini di consentire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti costituenti reato in una circostanza che non rendeva facile l'accertamento della loro identità. L'articolo 5 riguarda la violazione del regolamento sull'utilizzabilità degli impianti. L'articolo 6 introduce misure di prevenzione (anche misure di prevenzione antimafia ) sia personali che patrimoniali. L'articolo 7 concerne

virtuose. L'articolo 9 concerne prescrizioni per le società che organizzano le competizioni del gioco del calcio. Quindi, esso riguarda piuttosto la vendita dei biglietti; al riguardo, sono state introdotte nuove disposizioni che rendano assai più stringenti ed efficaci

l'adeguamento degli impianti. Si introducono misure assai semplificatorie e acceleratorie per ottenere i permessi necessari per adeguare gli impianti alle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 11 mira a promuovere programmi e cultura nuovi

fruttuoso anche quel lavoro emendativo che si è cercato di svolgere in seguito. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti i senatori che hanno partecipato a questo lavoro perché è stato assai rapido e facile conseguire un clima molto costruttivo all'interno delle Commissioni. Il lavoro emendativo svolto credo che sia stato importante. È stato possibile trarre da tutte le questioni che sono state affacciate delle sintesi assai significative. Il testo è stato largamente migliorato, a mio avviso, con il contributo di tutti. Credo che una testimonianza di questo lavoro sia anche il fatto che oggi io e il collega Di Lello Finuoli siamo qui a rappresentare questo provvedimento con il mandato favorevole unanime

l'articolo 7 abbiamo ritenuto di convenire, sulla base di una proposta formulata dai colleghi D'Onofrio ed Eufemi, che la resistenza a pubblico ufficiale, reato di mero pericolo, potesse essere sostituita con una misura assai più impegnativa di innalzare significativamente le pene per coloro che provocano lesioni gravi o gravissime nei confronti di pubblici ufficiali in occasione di eventi che concernono l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lepene che sono state individuate configurano un'ipotesi autonoma di reato e portano le lesioni gravi nei confronti di pubblici ufficiali in occasione di attività di ordine e sicurezza pubblica

Questo perché il monito deve essere serio, soprattutto quando si evidenzia un fatto oggettivo come quello non soltanto di avere attentato alla vita della persona, ma addirittura di averne provocato conseguenze dannose attraverso la produzione di fatti lesivi della propria integrità personale. Un'altra misura che abbiamo voluto adottare di comune accordo dinanzi a molti emendamenti presentati da quasi tutti colleghi, e molti di questi dal senatore Castelli, è stata di ritenere di non dover affrontare qui nel merito il tema degli *stewards*

di dover prevedere con un emendamento che debba essere il Ministro dell'interno a promuovere un decreto che regoli la selezione, il reclutamento, la formazione e le modalità di collaborazione con le Forze di polizia di questo personale anche perché non tutti potrebbero essere impiegati in attività che potrebbero richiedere una collaborazione con le Forze di polizia. Quindi, ci è sembrato opportuno che un decreto del Ministro competente

tratta certamente di un passo in avanti rispetto al cosiddetto decreto Pisanu perché prevede, in una materia come quella in esame, il pieno coinvolgimento del Parlamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono poche le questioni che residuano e meritano di essere citate singolarmente. Mi sono voluto limitare a quelle due che hanno occupato

Abbiamo redatto un provvedimento con lo spirito comune di perseguire davvero il bene di tutti senza guardare a maggioranza o a opposizione, a singoli partiti o a singoli senatori. Tutti hanno collaborato per rendere più efficace e migliore il testo.

fatta dal senatore Sinisi non mi rimane che aggiungere qualche notazione. Devo però convenire con il collega Boccia sul c'è una difficoltà nella lettura del testo perché sono riportati tutti gli emendamenti, e quindi una lettura di quello su cui abbiamo avuto un parere concorde in Commissione può essere fatta soltanto seguendo gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite. Dobbiamo anche dare atto agli Uffici

che fosse la semplice riproposizione di tutti gli emendamenti, più quelli approvati dalle Commissioni riunite. Mi vorrei soffermare su alcuni punti.

introdotte in questo decreto. In Commissione non si è raggiunto un accordo; c'è stato un ampio dibattito, il Governo ha mantenuto la sua posizione di tener fermo l'articolo 6. Devo dire - per amore della verità che la Commissione si è divisa su due pareri: una parte era d'accordo

L'orientamento principale e prevalente è stato proprio quest'ultimo. non sia opportuno inserire in questo decreto le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste per le organizzazioni mafiose ed altro, proprio perché non è necessario. A parte il fatto che in Commissione antimafia cominceremo a studiare un testo unico che razionalizzi questo tema, credo che non sia necessario inserirlo, perché se questi Gruppi

quindi rimesso alla discussione dell'Aula questo tema; l'Aula è sovrana e deciderà. Personalmente, per la mia esperienza e per il lavoro che facciamo anche in Commissione antimafia, credo sia inutile. Per il resto il decreto è un buon decreto, nel senso che si sovrappone al decreto Pisanu, però lo migliora in molte parti, lo rende un po' più razionale e accoglie anche suggerimenti venuti dalle Forze di polizia. Per esempio le Forze di polizia ci hanno detto con molta chiarezza che questo sistema del biglietto nominativo,

esibendo due biglietti, uno intestato a Francesco Baracca e un altro a Gaetano Bresci: credo che in qualsiasi stadio, almeno Gaetano Bresci non verrebbe fatto entrare. Tuttavia, ripeto, questo commissario di polizia

una cosa utile e un'altra cosa inquietante, come ho già riferito in Commissione, cioè che la settimana dopo l'entrata in vigore di questo decreto, allo stadio di Bari

Per il resto non ho altro da aggiungere, credo che il lavoro che abbiamo svolto in Commissione - come già detto dal collega Sinisi - sia stato ottimo; si è raggiunta l'unanimità almeno sui punti che presentiamo come frutto del lavoro delle Commissione riunite e, ripeto, tranne l'articolo 6, in realtà questo è un lavoro che

a una rapida votazione. Spero solo che - come era stato sollecitato dal collega Antonio Boccia e come ha saggiamente suggerito il Presidente

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, interviene in maniera urgente in una situazione di fatto grave che stava degenerando vieppiù. Quello che era un gioco, uno splendido spettacolo (per qualcuno il migliore del mondo), si è trasformato oggi in Italia in qualcosa di molto diverso, qualcosa di patologico, in un problema anche grave di ordine pubblico. Era ed è evidente, perciò, la necessità di porre rimedio o, almeno, il tentativo di porre rimedio, a tale stato di cose, anche se, a mio parere, già prima del decreto-legge n. 8 del 2007, il problema non era da considerarsi soprattutto sotto il profilo normativo, perché il sistema delle norme già c'era, sia da un punto di vista sostanziale che procedurale. Mi limito a citare gli istituti dell'arresto in flagranza, del rito per direttissima e l'esistenza di pene anche gravi. La normativa vigente in materia era già repressiva; bastava applicarla. Questa è stata la principale manchevolezza successivamente all'entrata in vigore del decreto Pisanu. Peraltro, nella grave situazione venutasi a creare particolarmente dopo i gravissimi episodi di Catania, era necessario e indispensabile dare un segnale politico forte di attenzione, che da parte del Governo, sia del Parlamento. Noi non partiamo, legislativamente parlando, da zero: già esistono le norme introdotte con il cosiddetto decreto Pisanu e su quella strada, positivamente segnata, ci dobbiamo inserire anche ora con il nuovo decreto-legge. presente decreto n. 8 del 2007 introduce delle correzioni, delle integrazioni, dei ritocchi a quell'impianto normativo e fornisce delle indicazioni nuove che, in prospettiva, dovranno condurre a ipotesi risolutive; ma soprattutto vuole dire chiaro e forte che non è accettabile che il gioco del calcio da spettacolo si sia trasformato in un problema di sicurezza. Le soluzioni prospettate concretamente dal decreto-legge al nostro esame sono del tutto positive, soprattutto per i seguenti aspetti. Innanzitutto, si è intervenuti per rendere concreta e applicata la precedente normativa del decreto Pisanu in materia di sicurezza degli stadi, normativa rimasta colpevolmente inapplicata dopo l'entrata in vigore di quel decreto. luogo, è stato in maniera precisa e più corretta regolamentata la questione relativa al divieto di acceso negli stadi, tale divieto, in particolare, diventa preventivo (così si parla di DASPO). C'è un ragionato inasprimento delle pene, non assurdo, non slegato dal sistema, soprattutto dopo le correzioni che sono state apportate in sede di Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali,

Con gli emendamenti e le discussioni avvenute in sede di Commissioni riunite si è adeguatamente riconsiderata la questione della violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte in sede di audizione dai rappresentanti della Polizia di Stato e dai rappresentanti sindacali di polizia. di polizia. L'adeguamento degli stadi, già previsto dal decreto Pisanu, viene posto a carico delle società sportive utilizzatrici degli impianti. Sono state poi inserite norme utili e importanti anche da un punto di vista formativo, sportivo e culturale, a partire dall'articolo 11, e con le correzioni e gli inserimenti effettuati in sede di Commissioni riunite. E' chiaro che, come per ogni legge, non tutto è stato previsto e non tutti i problemi sono stati risolti. Cito, ad esempio, tre questioni: la prima è quella relativa agli *steward*, gli organi di vigilanza privata, questione che dovrà essere certamente ripresa in esame, in un ambito peraltro più vasto; la seconda questione, per certi versi collegata alla prima, è quella relativa alla proprietà degli impianti sportivi; la terza questione è quella relativa alle sanzioni nei confronti delle società. Se esistono, come sicuramente esistono, alle volte rapporti oscuri e pericolosi tra alcune società e alcuni gruppi di tifosi, è evidente che vanno meglio individuati tali contatti, che vanno meglio individuate le strade per accertare tali contatti e rapporti e vanno previste sanzioni più adeguate. Rischia di non risolvere nulla la sola previsione di una sanzione amministrativa, tra l'altro di importo tutto sommato limitato, soprattutto per le società maggiori. Andrà studiata e approfondita la possibilità di intervenire con sanzioni più gravi e adeguate nei confronti delle società, quali ad esempio la penalizzazione in punti o la limitazione delle trasmissioni via TV. In conclusione, ritengo però che il segnale politico che è stato dato e deve essere dato al mondo dello sport, e del calcio in particolare, deve essere chiaro e forte. Non è questo un settore del quale ci dobbiamo o possiamo disinteressare. Per evitare l'aggravarsi di situazioni di pericolo e di emergenza di ordine pubblico, ben venga questo decreto che con convinzione va approvato senza alcun indugio. È certamente molto positivo che alla miglior formulazione di questo decreto-legge abbiano partecipato senatori sia della maggioranza che dell'opposizione. È questo un ulteriore segnale positivo che viene dato al Paese, nella consapevolezza che, di fronte a problemi di sicurezza così delicati e rilevanti, è fondamentale agire con uno spirito comune e unitario. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà. Signor Presidente del Senato, signor rappresentante del Governo, colleghi, certamente questo provvedimento ha un grande valore

si registra un fatto positivo: non si parla da parte della maggioranza di discontinuità rispetto a provvedimenti precedenti, bensì di assoluta continuità. Questo, forse, è un segno dei tempi o del cambiamento dei tempi che stiamo vivendo. Finora su ogni provvedimento la maggioranza aveva cercato di segnare la completa discontinuità rispetto a ciò che il precedente Governo aveva fatto, mentre in questo caso si è riconosciuto che il decreto Pisanu è stato assolutamente positivo, anche se in parte non applicato. Questo provvedimento, su cui ci si è molto soffermati in Commissione, che porta ad una serie di aggravamenti di pene e di aumenti di divieti, coglie

rapporto «delittuoso» tra i *fan*, gli ultras delle società sportive e in generale il resto dei tifosi, il mondo del calcio e la passione per esso. Oggi

non era più possibile accettarlo; era necessario rompere, attraverso questo provvedimento, quel nesso, che talvolta ha generato questa violenza, tra le società e gli ultras. È noto che le società hanno sempre fornito agli ultras biglietti gratis, servizi; hanno fatto gestire loro il *merchandising.* Questo ha creato in molte occasioni delle situazioni di pericolosità che poi si sono trasformate evidentemente in incidenti molto pesanti. La vicenda di Catania, comunque da, tutti gli analisti è stata interpretata non solo come una vicenda di natura sportiva, bensì come una vicenda legata al disagio sociale di quella città, ad una avversione pesantissima nei confronti della e l'evento sportivo, la partita Catania-Palermo ha assunto altri significati, che andavano al di là della vicenda sportiva. Sono però convinto che non solo con la repressione, con queste misure

ha consentito in quindici giorni a molte società e a molti Comuni di dar corso all'utilizzazione di quelle attrezzature (tornelli, fotocamere, *metal detector*, *metal detector*, videocamere) e tutte quelle strutture che invece sembrava fosse difficile recuperare. Abbiamo fatto quel grande capolavoro che tutti sanno: abbiamo fatto aumentare del cinquanta per cento il costo dei tornelli perché ve ne erano pochi in circolazione; sta di fatto, però,

sono convinto che con queste misure repressive non si risolverà la crisi del calcio. Come è noto, solo nell'ultimo anno vi è stata una diminuzione di spettatori negli stadi italiani parlo soprattutto degli stadi dove giocano squadre professioniste - del 30 per cento: la vicenda di Calciopoli, la violenza, altri fenomeni che si sono venuti ad ingenerare creato sostanzialmente una fortissima disaffezione nei confronti di questo grandissimo fenomeno sportivo. In secondo luogo, bisogna tenere conto che negli ultimi dieci-quindici anni, con l'ingresso delle *pay-tv*, è cambiata sostanzialmente l'impostazione, la struttura dei bilanci, il modo di fare calcio. È diventato un più che sportivo, di grande rilievo economico. Da questo bisogna partire per cambiare la qualità dell'impostazione di tutta la vicenda calcio. Sono convinto che se dopo questo provvedimento non vi sarà un provvedimento quadro che affronti in particolare particolare la questione stadi e la loro gestione, (questione che andrà affrontata non solo con provvedimenti di natura parlamentare, bensì anche d'intesa con gli enti locali che in molti casi sono proprietari degli stadi) non si riuscirà a risolvere questa vicenda. Sono convinto che, come ormai sta avvenendo in tutti i Paesi occidentali (dall'Olanda alla Spagna all'Inghilterra), gli stadi debbano essere privatizzati e la gestione della sicurezza all'interno degli stadi debba essere di completa responsabilità delle società. Oggi le società di calcio, soprattutto con gli introiti delle *pay-tv*, hanno una enormità di risorse finanziarie; le destinano in modo assolutamente marginale alla gestione della sicurezza, ma essenzialmente all'acquisto di calciatori, al pagamento degli ingaggi. Dobbiamo costruire un modello, come si è riusciti a fare in altre parti di questa Europa, in cui le società sono proprietarie, gestiscono gli stadi, si assumono le responsabilità su chi entra, gestiscono l'ordine pubblico al loro interno e non sta più succedendo nessun fatto delittuoso.

se uno è un delinquente e vuole usare il fenomeno sportivo del calcio per altre ragioni, non gli è consentito di entrare. Le società svolgono una funzione di filtro, che blocca tutto. Allora, la mia opinione è che questo provvedimento è positivo ed importantissimo; però dopo questo provvedimento,

In Italia siamo in presenza di stadi assolutamente obsoleti. Quelli realizzati per i Campionati del mondo del 1990 non sono più utilizzabili rispetto alle esigenze attuali, sono stadi con piste di atletica che vanno assolutamente modernizzati. Se prevederemo qualche forma di incentivo per la loro privatizzazione o per la realizzazione di nuovi impianti e affideremo la gestione totale della responsabilità dell'ingresso negli stadi alle società questa vicenda si chiuderà definitivamente. Esprimo pertanto apprezzamento per il provvedimento, però bisognerà fare uno sforzo ulteriore, altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno ad avere tante Bari, come ha indicato il relatore, perché in Italia si fanno le leggi ma poi non si rispettano e i problemi tornano a proporsi. Dobbiamo quindi evitare che ci siano tante vicende come quelle accadute in queste ultime settimane a Bari e per questo ci vuole una svolta radicale.

il lavoro serio e rigoroso che è stato svolto dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia ha consentito di apprezzare la proposta del Governo, che credo sarà sicuramente votata, così come peraltro in

Galimberti parte dalla considerazione che la mitezza delle pene, peraltro spesso inapplicate, porta a ripetere con la cadenza del rito ciò che all'inizio era solo un fatto isolato.

latente nell'inconscio individuale di ciascuno di noi, diventa manifesta nell'inconscio collettivo di massa, dove la responsabilità individuale diventa difficile da identificare e l'impunità generale diventa un salvacondotto per gesti più esecrati e senza motivazione, perché la violenza assoluta è autosufficiente. Di qui, conclude Galimberti, la necessità di «interrompere il rito», la ritualità settimanale di esercizio di violenza. Interrompere il rito, quindi sospendere le partite, sospendere le attività sportive. Credo invece che l'interruzione del rito segnata non solo dall'interruzione della partita ma dall'intervento forte, deciso e rigoroso della legalità. Occorre ristabilire il principio di legalità. Di fronte a quanto è accaduto a Catania ho ascoltato l'intelligenza degli interventi dei rappresentanti del CONI, della Federazione, del mondo sportivo e anche della politica, del Parlamento e del Governo;

Di fronte al corpo straziato dell'agente di Polizia, quel procuratore aggiunto si è permesso di dire che avrebbe sequestrato lo stadio, quando lì non era avvenuto alcunché, perché le vicende erano accadute fuori. Dove vi erano le prove di quanto accaduto, il giorno dopo è stato consentito che si tenesse un mercato: quindi, le prove sono andate disperse. Domando ancora:

Non conosco processi seri; non ho visto un'applicazione piena del nostro sistema penale nei confronti di costoro. Basta una manifestazione sindacale o studentesca per arrivare, magari, ad arresti per reati effettivamente contestabili;

ma il nostro codice è pieno di reati inapplicati nei confronti di costoro. Vedendo quanto accaduto a Catania, avrei potuto elencare decine di reati commessi: non sono stati fermati nel momento in cui quella violenza veniva perpetrata? Perché non sono stati fermati e arrestati? Questo era il segno vero

appunto, fermare i violenti e, la mattina dopo, portarli sul banco degli imputati, processarli e condannarli se colpevoli, con tutte le dovute garanzie: questa la risposta che lo Stato avrebbe dovuto dare e non ha dato.

non sono sufficienti. Occorre togliere quest'area di impunità nei confronti dei violenti; bisogna ritornare ad un'applicazione seria, rigorosa delle norme che già vi sono. Quelle associazioni sportive assomigliano molto ad un'associazione per delinquere, eppure mai è stato contestato l'articolo 416 del nostro codice

si manifestino atti di violenza e di illegalità, come quelli che avvengono settimanalmente negli stadi del nostro Paese. Ha dunque ragione Galimberti: occorre interrompere quel rito; non basta, però, sospendere la partita o impedire che i violenti entrino nello stadio: occorre che chi è violento paghi per i suoi atti insensati, per la sua condotta illegale, così come qualsiasi altro cittadino. I magistrati,

(non è difficile, infatti, trovare sostituti procuratori allo stadio, che il lunedì rimangono silenti). Occorre che la magistratura svolga gli atti doverosi che deve compiere, perché l'azione penale è obbligatoria.

Stato forse l'aggressione di Catania non ci sarebbe stata e quel povero agente oggi sarebbe ancora con la sua famiglia. Naturalmente, approveremo

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io colgo come un elemento importante la rapidità, nonostante le fibrillazioni di questa fase, con cui affrontiamo questo delicato provvedimento. È il segno di come sia forte la consapevolezza nel Governo, e credo in tutto l'arco costituzionale, della vera e propria emergenza che ci troviamo a discutere. conversione che oggi siamo chiamati a votare assolviamo ad un primo impegno che, con parole unanimi, quest'Assemblea aveva preso all'indomani dell'omicidio dell'ispettore Raciti. Non siamo di fronte a una risposta emotiva di corto respiro ma all'affermazione netta che non esistono nel Paese luoghi dove le regole della convivenza sono sospese. Negli stadi non vige l'extra territorialità; era un segnale necessario e urgente ma siamo tutti consapevoli che non è sufficiente. Il provvedimento interviene innanzi tutto sul lato della repressione. Per me le direttrici sono tre e ora servono interventi forti tanto sul terreno della prevenzione quanto su quello dell'azione sociale. Dobbiamo essere capaci di prosciugare il contesto culturale entro cui si formano i violenti; serve un percorso coraggioso e partecipato che consenta al nostro calcio una piena assunzione di responsabilità. L'autonomia dello sport è un valore che nessuno ha mai messo in discussione ma l'autonomia ha anche un prezzo che si chiama responsabilità. Dopo questo importante intervento, servono allora ulteriori provvedimenti, a partire dalla gestione degli stadi per arrivare alla responsabilizzazione, appunto, delle società. Spero che con pari celerità e puntualità sapremo completare un disegno complessivo che ci consenta di dare risposte strutturali capaci di sconfiggere la violenza legata agli eventi sportivi. Lo dobbiamo fare con la consapevolezza di cosa sia lo sport nel nostro Paese, grande fenomeno sociale che coinvolge milioni di cittadini - siano essi atleti, tifosi, amatori - e non vorremmo che passasse una semplificazione assai grave, quella per cui la moltitudine dei cittadini sia spesso connivente con i violenti e i facinorosi. Nel mondo dello sport e anche nel tifo ci sono valori e passioni che possono essere il più forte antidoto contro la violenza; sono quei valori di disciplina e rigore che l'attività sportiva spesso sa insegnare. Nel merito del provvedimento, non vorremmo che la scelta di giocare a porte chiuse per gli stadi fuori norma nascondesse un intervento che credo vada sottolineato: il rafforzamento del divieto di rapporti economici tra società e tifo violento, che è cosa diversa dal tifo organizzato. Vietare con forza e rigore le connivenze tra società e tifosi è un passaggio determinante per la costruzione di un diverso modello di sport, e particolarmente importante per il calcio, così come un rafforzamento della nominatività dei biglietti diventa un altro passaggio cruciale. Sono certo che queste nuove procedure di controllo verranno anche adeguatamente monitorate. Un ulteriore percorso dovrebbe essere, almeno in via sperimentale, l'automazione del tracciamento nell'area degli stadi, scelta che non sarebbe in contrasto con la nostra normativa sulla *privacy*. Dopo il voto della prossima settimana per la conversione in legge del decreto in questione, abbiamo la responsabilità di dare continuità, come legislatori e come istituzioni, a questa battaglia. La scelta contenuta nell'emendamento del Governo che prevede interventi nelle scuole è un primo forte segnale, per il quale esprimiamo vivo apprezzamento e forte soddisfazione. Ma è un segnale che va rafforzato: i valori dello sport non si raccontano, ma si praticano con il sudore nei campi di calcio e nelle palestre. Per questo speriamo di incontrare la sensibilità di tutte le forze e di tutte le istituzioni a proposito dell'urgenza di un piano organico per le palestre scolastiche

potersi formare lungo il percorso educativo. Costruire un disegno complessivo è quindi il nostro intendimento, e questo provvedimento rappresenta il primo tassello. Ma per farlo dobbiamo avere un'idea chiara e condivisa. Un primo punto di questo disegno è che nello sport i valori devono rimanere più forti del mercato e anche del profitto: un calcio organizzato in funzione delle televisioni è uno spettacolo onestamente distorto e desolante. Dobbiamo correggere con forza questa tendenza. II CONI e la FIGC innanzitutto devono riaffermare con forza che il calcio è uno sport e non un mercato. Ma questo è un dovere di tutte le istituzioni, ciascuna con il proprio ruolo. è rappresentato dalla consapevolezza che la partecipazione è la prima leva di riforma dello sport: abbiamo troppo spesso visto le componenti sportive l'una contro l'altra, e questo è inaccettabile. La recente approvazione dello statuto della FIGC è un segnale positivo che va incoraggiato. Ma serve che questa consapevolezza sia anche delle istituzioni. Noi abbiamo l'ambizione di poter frequentare stadi dove non sia pensabile un comportamento violento, dove l'intimidazione non sia una prassi accettata, dove la bellezza del gesto sportivo sia la vera protagonista, e non gli assalti tra le tifoserie o contro la polizia. Questo è possibile solo se rafforzeremo il tifo organizzato e corretto, se lo accetteremo come un interlocutore. Responsabilizzando tutte le componenti, e rifiutando la semplificazione per cui i tifosi sono una folla indistinta, avremo uno strumento forte ed efficace contro la violenza. In questa direzione va un mio emendamento che cerca di esplicitare il potere dei prefetti e di convocare periodici tavoli di lavoro con le componenti del calcio. Sarebbe uno strumento utile che ci aiuterebbe a dividere i violenti dai tifosi.

una condivisione di fondo e quindi potremo esporre considerazioni che non vogliono essere polemiche o di contrapposizione politica. politica. Il Governo precedente nella scorsa legislatura si è occupato più volte del tema della violenza negli stadi. Viene sempre evocato il decreto Pisanu, ma in realtà

allo stadio, sulle tribune o anche per strada. È chiaro che la Polizia assume atteggiamenti prudenti ma, con i mezzi mediatici a disposizione in questi tempi, è possibile filmare queste persone, individuarle, identificarle nelle ore successive.

devo ricordare con rammarico - e lo dico perché poi riprenderò il tema in coda al mio intervento - che quella norma venne bocciata dal Parlamento

non soltanto di prevenzione ma anche di intervento successivo per identificare chi si macchia di questi che sono veri e propri delitti. Come dicevo, si tratta anche di un elemento di prevenzione, perché il facinoroso che prima di oggi si sentiva

del Regno Unito, dove esisteva la piaga degli *hooligans* che oggi, se non del tutto eliminata, è stata comunque in larga parte circoscritta. Qualcuno ha qui evocato le grida manzoniane. Credo che questo sia il punto fondamentale. A mio giudizio, la battaglia che dobbiamo portare avanti, e che non è stata sufficientemente fatta, è sul piano culturale. Per troppo tempo si è tollerato in questione agissero indisturbate all'interno, tra l'altro, di una politica della tolleranza molto più vasta. Ricordo che

con il nome che hanno, cioè sediziosi quandanche non dei criminali, che vanno colpiti con gli strumenti che lo Stato ha per colpire gli stessi criminali. Lasciatemi segnalare - lo faccio senza polemica -

tutti i provvedimenti che adotteremo in questa Aula saranno vani. Termino con un riferimento a quanto sostenuto dal collega Calvi sugli interventi della magistratura. Il mancato intervento della magistratura è figlio proprio di questa cultura,

riteniamo giusto ed opportuno il decreto-legge dell'8 febbraio 2007, come riteniamo giuste ed opportune le riflessioni del ministro Amato sulla necessità di fermare la violenza negli stadi. Integrare e migliorare la normativa di contrasto alla violenza varata nella precedente legislatura dal ministro Pisanu dopo l'omicidio dell'ispettore di polizia Raciti è giusto, opportuno e doveroso.

Questo decreto indica strumenti di prevenzione che modulano l'organizzazione di manifestazioni sportive di calcio, l'adeguamento degli impianti sportivi senza più deroghe, la limitazione della vendita dei biglietti alla tifoseria della squadra ospite, la regolazione degli spostamenti collettivi dei tifosi, l'inasprimento delle misure interdittive per i tifosi violenti e l'ulteriore inasprimento delle pene pecuniarie e detentive, la flagranza differita del reato fino a 48 ore dal fatto nei confronti di autori precisi responsabili di minaccia, resistenza, violenza e attività offensive e aggressive verso le forze dell'ordine e civili, la limitazione nei confronti delle società di calcio di sostenere e agevolare il tifo organizzato, un'attività volta a migliorare e favorire l'adeguamento tecnico degli impianti soggetti a misure di sicurezza secondo i parametri dei decreti Pisanu. L'UDC sul provvedimento ha dato un contributo costruttivo e si è mossa su tre filoni: la tutela delle forze dell'ordine, la regolamentazione della vendita dei biglietti, migliorando il testo del Governo soprattutto per la parte non prevista della vendita dei biglietti in caso di *derby* con la riproposizione in Aula, per garbo e trasparenza istituzionale, di un ordine del giorno già approvato in Commissione, e la promozione della cultura dello sport su ampio spettro di opportunità.

soprattutto in merito all'uso degli addetti alla sicurezza non appartenenti alle forze dell'ordine. Ci sono implicazioni di carattere giuridico che meritano un approfondimento tecnico per i risvolti di carattere civile e penale. Abbiamo perciò rimesso ad una delega legislativa un'articolazione puntuale e precisa sugli istituti giuridici più opportuni da applicare. Si tratta quindi di un ulteriore giro di vite. Salvo qualche eccezione, tutte le società sportive aderenti alla Lega calcio hanno accolto favorevolmente le ulteriori misure di sicurezza imposte dal Governo. Anche il mondo politico ha reagito positivamente, salvo il presidente del Club Roma Montecitorio. L'intervista di questo autorevole Vice Ministro alla stampa dello scorso 5 febbraio è un capolavoro di diseducazione alla legalità. A parte il cattivo gusto di criticare il proprio Governo, al quale c'ha abituato questa maggioranza di centro-sinistra, si dà voce a quella cultura deviata che vede nelle forze dell'ordine un nemico da colpire. Lavicenda dell'omicidio Raciti è infatti rivelatrice di questo tipo di cultura. Non solo i dati del Ministero dell'interno indicano che da quando è in vigore la legge n. 210 del 2005 i feriti negli incontri di calcio sono diminuiti del 7 per cento, ma anche che i feriti sono stati limitati solo sul fronte dei tifosi perché tra le forze dell'ordine sono aumentati del 42 passando da 142 del 2005 a 202 del 2006. Nella stessa partita Catania-Palermo tra i 90 feriti registrati 20 agenti sono stati ricoverati in condizioni preoccupanti, uno in fin di vita e uno, Filippo Raciti, è deceduto. All'indomani di questa tragedia a Livorno è apparsa la scritta: «uno in meno». A Genova invece la vittima è stata assimilata alla vendetta degli ACAB, acronimo di *all *all cops are bastards,* cioè tutti i poliziotti sono bastardi, nati sulle ceneri del G8 per ricordare la morte di Carlo Giuliani. È su questo aspetto dell'ostilità verso le forze dell'ordine che intendo concentrare l'attenzione perché rivelatore di un sentimento violento, ribelle, cattivo verso il prossimo e la società. Il poliziotto è l'ordine. È lo schema mentale in cui si realizza un'organizzazione di esseri umani razionale, ordinata, armonica. Contestare e distruggere questo schema per sostituirne un altro è comprensibile anche se non condivisibile, ma contestare e distruggere con logiche del noto film «Arancia meccanica» non solo non è condivisibile ma è incomprensibile. Una gioventù violenta, rabbiosa, senza schemi, senza futuro, senza idee non merita né comprensione né tolleranza. Va repressa e basta. pene severe e carcere duro, non solo per il calcio ma per ogni tipo di violenza e in ogni occasione in cui essa si manifesti: pirati della strada che ammazzano e fuggono; diverbi di condominio che finiscono a coltellate, fucilate o addirittura in stragi, come quella di Erba. Fin qui si potrebbe affermare che siamo nella fisiologia di un sistema sociale, ma non ci siamo più quando il bullismo nelle scuole diventa normale; quando i vandalismi nelle scuole e nei centri storici diventano fenomeni accettati come espressione del disagio sociale e ci si rassegna; quando è normale che su Internet si trasmettano video di pestaggi ad handicappati e ad extracomunitari ovvero violenze sessuali a minorenni e vengano accettati come fenomeni goliardici che una certa sociologia è arrivata a comprendere e a difendere. Ho ancora in mente l'inchiesta de «Il Messaggero» sull'uso della cocaina diventato non solo diffuso, ma anche un requisito nobile di diversità che pervade i ceti sociali più abbienti ed anche quelli popolari. Non dimentichiamoci, poi, la campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere e l'uso dello spinello come se fosse un pacchetto di Marlboro. Potremmo proseguire osservando le stragi del sabato sera conseguenti alla moda dello sballo, all'uso dell'alcool come atteggiamento di maturità degli adolescenti che sta rovinando migliaia di giovani. Ci chiediamo il motivo di questa deriva: crisi della famiglia, crisi della scuola, crisi delle agenzie educative o crisi di valori forti? Probabilmente si tratta di tutto un po', ma la stigmate della crisi di identità dei giovani è data dalla sopraffazione di modelli di vita imposti dal consumismo televisivo e cinematografico. C'è un plagio mediatico, a cominciare dalla televisione di Stato, che propone modelli di vita violenti e trasgressivi, che deviano e corrompono la mente e la personalità dei giovani. Il Ministero per le politiche giovanili deve interrogarsi su questo tema. Si tratta di capire dove i diritti personali e i diritti di libertà personale si possono comporre tra loro perché la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. I giovani devono essere protetti. L'UDC, sulla droga, sulle stragi del sabato sera, sull'uso dell'alcool, sulla stigmatizzazione del bullismo, ha fatto sentire più volte forte e chiara la propria voce per proteggere, aiutare e sostenere i giovani. I giovani sono il nostro futuro, ma una cultura permissiva, lassista ed indifferente ci ha finora sopraffatto e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Cultura della legalità nelle scuole, nella famiglia, nello sport ed in tutte le agenzie educative è l'imperativo categorico della politica. La severità ed il rigore a tutti i livelli rappresentano la cultura da affermare se vogliamo salvare i giovani e la società italiana nel suo immediato futuro. Questa è la linea politica dell'UDC ripetuta in tutte le sedi e che sarà ribadita fino alla noia perché le leggi ci sono e devono essere applicate. Ha ragione il collegaCalvi quando afferma che non occorrono leggi speciali, ma bisogna applicare quelle esistenti. Non si può pensare per ogni emergenza a leggi di emergenza. Difendiamo un Paese normale. Per tale motivo, voteremo a favore del provvedimento in esame e di altri che avranno lo stesso spirito per il bene dei nostri giovani e della società italiana.

credo - anzi sono convinta - che l'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania non sia soltanto la più recente e grave manifestazione della violenza,

è un atto, pare, deliberato, rivolto contro un pubblico ufficiale di polizia, impegnato personalmente e direttamente nel nel contrastare la violenza negli stadi; per l'età bassa, sempre più giovane, di chi ha commesso questo atto; per il contesto in cui è avvenuto e gli intrecci con forme organizzate di estremismo politico, razzista, di destra, e per il contesto sociale culturale, tanto che anche nel nostro provvedimento si è pensato bene di far riferimento a norme che riguardano la mafia. la mafia. Ciò ha motivato il Governo a razionalizzare e migliorare, in parte integrare, le norme che già c'erano, quelle del decreto Pisanu,

L'unanimità che abbiamo raggiunto non era affatto ovvia né scontata; potevamo ritenere ovvio che non ci fossero divisioni politiche sulla necessità di contrastare la violenza negli stadi, meno ovvie le analisi su questo e le risposte da dare. Abbiamo lavorato a rafforzare quanto già era presente nell'impianto del decreto: la prevenzione della violenza. Prevenzione non solo in senso securitario della polizia e della magistratura rispetto a comportamenti che possono divenire reati, ma prevenzione in senso più strutturale: dalle norme sugli impianti, cioè sui luoghi, sulle strutture persino fisiche, i luoghi materiali in cui avvengono le manifestazioni, a quelle su che cosa è diventato il calcio in questo Paese, le società, i rapporti tra le società e le consorterie dei tifosi e degli ultras. Quindi, rafforzare la responsabilità delle società rispetto a simili fenomeni, prevedere sanzioni nei loro confronti e interrompere, spezzare appunto, quei legami attraverso i quali non solo favoriscono, ma spesso addirittura organizzano, promuovono e sovvenzionano organizzazioni che sono quelle che poi portano alla esplosione della violenza negli stadi. Non credo quello che pensa il senatore Saro e che altri hanno detto, vale a dire che la privatizzazione sia l'unica risposta. Questa è una delle tante scorciatoie che forse dovremmo evitare nel porre il problema di una diversa responsabilità delle società e di un diverso ruolo delle società sportive per modificare e intervenire più in profondità nell'esercizio

pare già qualcosa di fortemente privatistico, che non possa essere quindi affrontato e risolto dicendo privatizziamo ulteriormente, fino agli stadi. Prevenzione, anche e non solo strutturale; l'articolo 11 si propone di intervenire sulla cultura, nelle scuole e nella società, in senso più lato; cultura civica, sportiva, politica, visto che ogni volta che c'è un problema di violenza, c'è un problema di democrazia. Alcuni colleghi si sono avventurati anche in letture sociologiche, antropologiche o in semplificazioni politiche che, francamente, mi sembrano fuori luogo. Non mi metto su questa strada. Voglio solo ricordare che analisi e studi seri di antropologia sociale e politica sullo sport, da un lato, riconoscono che la competizione ha sempre in sé un elemento di violenza (l'agonismo che deriva dalla cultura greca) greca) perché, appunto, contrapposizione e riproduzione dello schema vincitori e vinti. Se questo non vi dice niente sulla cultura politica che sta prevalendo, non solo in questo Paese, ma nel mondo, sulla militarizzazione e sulla risoluzione

manca la prevenzione, quell'aspetto che le norme penali spesso introducono. Applicare le norme esistenti è un modo per prevenire che comportamenti violenti e reati si riproducano.

che credo, in parte, dovremmo riprendere in sede di discussione degli emendamenti e che vorrei fosse oggetto di una riflessione più generale in quest'Aula: il ruolo delle pene, che può essere tanta parte del nostro lavoro. Non sottovaluto la gravità dei fenomeni di violenza. Non sottovaluto la responsabilità degli atti, né individuali, né, appunto, di società, di soggetti organizzati e collettivi. La mia domanda è un'altra: l'inasprimento delle pene ha davvero un'efficacia deterrente? Abbiamo alle spalle una storia, anche recente, di politica del diritto e del penale che ha portato i più autorevoli studiosi

la norma penale non è lo strumento più efficace per la prevenzione, perché prevenire vuol dire intervenire in altri modi, con altre politiche e altre norme, un altro uso del diritto e altri strumenti della politica che non siano soltanto la norma penale. Quindi, da questo punto di vista, ci dovremmo chiedere che cosa significhi riprodurre costantemente e regolarmente, dinanzi a ogni fenomeno da fronteggiare, quello che ho definito un riflesso quasi automatico. Sono fortemente contraria all'uso simbolico del penale, all'introduzione nel nostro ordinamento di leggi manifesto. Troppe ne abbiamo e ne ho fissa una in testa che che fa da paradigma: la legge n. 40 sulla procreazione assistita. Abbiamo pensato di risolvere fenomeni sociali rilevanti, che segnano la nostra società, con lo strumento del ricorso simbolico alla legge manifesto, tanto più negativa quando è legge penale. Non penso solo, come ha detto il senatore Di Lello, che l'articolo 6 non sia necessario.

Signor Presidente, Alleanza Nazionale ha manifestato interesse e attenzione alle comunicazioni del ministro Amato, che hanno fatto seguito ai fatti di Catania del 2 febbraio, e vorrebbe cercare una coerenza tra quelle dichiarazioni e le norme di questo decreto-legge. L'occasione della legge di conversione è importante per far sì che il Parlamento si assuma per intero la propria responsabilità sul fronte delle risposte che i problemi emersi così tragicamente a Catania, ma non soltanto a Catania, esigono. I problemi emersi negli ultimi anni sono problemi di rispetto delle regole, di applicazione delle sanzioni quando questo rispetto non c'è, di rispetto nei confronti di chi è chiamato a far applicare e ad applicare le sanzioni. Il rispetto delle regole chiama in causa anzitutto la piena, completa, immediata e chiara applicazione dei decreti attuativi della legge Pisanu, i quali hanno richiesto un lungo periodo di stesura che non è consistito in una perdita di tempo, ma nella ricerca di un percorso condiviso con tutti i soggetti chiamati in causa. Quei decreti si fondano su un protocollo sottoscritto non soltanto da parte dei Ministeri interessati alla loro applicazione, ma anche delle varie leghe (professionisti, semiprofessionisti, dilettanti, Federazione Italiana Giuoco Calcio, CONI

senza eccezioni e - mi permetto di aggiungere - senza rimpalli di responsabilità, come quelli che vi sono stati anche nelle ultime settimane tra società calcistiche e municipi su chi poi debba mettere mano al portafoglio per concretizzare quanto previsto nei decreti attuativi. L'alternativa è l'impedimento della manifestazione sportiva. Questa alternativa credo che

il percorso di addestramento e di formazione di coloro che saranno chiamati a svolgere attività di sicurezza all'interno degli impianti sportivi. Non è possibile affidarsi all'improvvisazione, né confidare per intero sulla capacità di selezione da parte di chi non ha questo compito, vale a dire le società sportive o i soggetti delegati dalle stesse. Ritengo

che disciplinerà le modalità di reclutamento, di addestramento e di formazione del personale della sicurezza interna ad impianti sportivi. I tempi non saranno rapidissimi. Viene indicato il limite dei 60 giorni per l'emanazione del decreto ministeriale, ma poiché questo decreto sarà inevitabilmente l'esito di un lavoro di consultazione con le associazioni di categoria, con gli addetti ai lavori, possiamo immaginare un tempo non straordinariamente maggiore, ma comunque maggiore. poi la necessità di un esame da parte del Parlamento così come questo articolo aggiuntivo prevede. I decreti applicativi della legge Pisanu sono invece immediatamente applicativi. Le partite non si giocano se non vi è il personale della sicurezza privata interno all'impianto sportivo. E come avviene oggi il reclutamento? Chi domenica prossima

la società sia condizionata dalle organizzazioni delle tifoserie, soprattutto da quelle più violente, anche per l'individuazione dei cosiddetti *stewards*? Per questo avevamo proposto un'ipotesi transitoria di requisiti analoghi, se non sovrapponibili, a quelli previsti per le guardie particolari giurate. Non ne facciamo un oggetto di scontro politico, ma semplicemente una proposta di riflessione ragionevole, per evitare che il periodo transitorio faccia sorgere dei problemi che andranno affrontati una volta che il sistema sarà reso definitivo. Certamente il riferimento che viene fatto nell'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge ai requisiti morali previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è, oltre che desueto, scarsamente concreto, evanescente. È necessario qualcosa di più. Noi manifestiamo soddisfazione sulla circostanza che il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO, nel lavoro delle Commissioni abbia conosciuto un significativo incremento nel minimo e nel massimo. Si è passati da un minimo di tre mesi e un massimo di tre anni ad un minimo di Siamo d'accordo con questo proprio perché riteniamo che - riprendo qualche intervento precedente - l'aumento della sanzione penale sia assolutamente inutile, ma l'incremento di una misura di prevenzione qual è il DASPO, sia pure di prevenzione atipica, sia ciò che più concretamente dissuade il violento, presente nell'impianto sportivo, dal tenere comportamenti coerenti con la propria visione del tifo. Siamo anche soddisfatti del fatto che, accogliendo alcune nostre proposte, il DASPO si possa applicare altresì nei confronti dei minori. Tutto ciò non significa incremento della sanzione penale, ma di una misura di prevenzione che ha un effetto limitato alla manifestazione sportiva e proprio per questo ancora più efficace. Vorremmo che questa misura fosse realmente applicabile. Per questo confidiamo nella circostanza che i lavori di Assemblea possano rendere i requisiti per l'emanazione della misura un po' più coerenti e più leggibili da parte dell'interprete, perché la norma, così come è stata scritta,

Non si riesce a capire se è un abbozzo di reato tentato o se è qualche altra cosa. Ma proprio perché esistono ancora delle incertezze, credo non si debba confidare sul lavoro ermeneutico della giurisprudenza, in particolare della Corte di cassazione, perché altrimenti ci ritroveremo con sentenze del giudice di legittimità il quale chiederà

le Forze di polizia. Va bene avere inserito questa nuova figura più seria per chi le colpisce in manifestazioni sportive; manca però, ed è oggetto di un nostro emendamento, un'ipotesi intermedia, cioè quella dell'oltraggio a pubblico ufficiale. Sappiamo bene che è stata eliminata dall'ordinamento qualche anno fa, ma la nostra non è una riproposizione secca di quella configurazione, bensì una riproposizione limitata agli interventi di ordine pubblico e di sicurezza, tesa a far sì che lo Stato, che attraverso la divisa di una persona in quel momento è esposto a particolare rischio, non attenda di essere raggiunto da una spranga perché intervenga l'autorità giudiziaria, ma anche quando per esempio c'è un dileggio grave, come uno sputo, si possa intervenire senza esigere dal poliziotto o dal carabiniere l'attivazione della querela,

tale decreto‑legge è frutto di un lavoro ampiamente condiviso, credo che per una volta tale pregiudiziale ideologica dovrebbe essere messa da parte. *(Applausi

è approdata in Aula sulla scia di un'onda emozionale provocata dagli ultimi gravissimi incidenti di Catania, che hanno costituito la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso che da lungo tempo andava riempiendosi con fenomeni sempre più frequenti di intolleranza, disordine e violenza. Dal confronto degli ultimi tre campionati calcistici risulta che gli arresti sono passati dall'8 al 35 per cento, le denunce dal 5 al 75 gli incidenti dal 28 al 97 per cento, i feriti dal 18 al 34 per cento. Il dato statistico generico riferito alla violenza negli stadi in quest'ultimo triennio calcistico ha registrato un forte incremento; infatti, dai 238 incidenti registrati nel 2000-2001 si è scesi ai 114 del 2001- 2002, per poi notare un'ascesa nel 2002-2003 con ben 290 episodi. Un dato significativo che può offrire ulteriore spunti di riflessione riguarda gli impianti sportivi; infatti, solo il 43 per cento risulta in regola, il 19 per cento sono inagibili, e di essi 10 sono considerati pericolosi. Il danno sociale di tale stato di fatto e di tali comportamenti è sotto gli occhi di tutti e non può essere trascurato, né permettere posizioni deboli. Una normale domenica allo stadio costa al Paese somme ingenti che vengono distolte da altre utilizzazioni. Il dato diventa ancora più allarmante se ci si sofferma ad analizzare il numero degli agenti delle forze dell'ordine utilizzati e il relativo costo sostenuto per ogni giornata di campionato. Questi i numeri: 7.760 uomini delle forze dell'ordine utilizzati dalla serie A alla serie C, di cui 5.040 della Polizia di Stato e 2.720 dell'Arma dei carabinieri. Per le prime venti giornate sono stati spesi 31,816 milioni di euro, di cui 569 per gli operatori feriti. Dati di questo genere, che ben servono ad inquadrare il fenomeno nel suo complesso, devono farci riflettere attentamente. Non è condivisibile la posizione di chi vede dietro tali fenomeni supposte ragioni giustificative di disagio sociale o povertà. Non dimentichiamo, infatti, che ogni volta che accadono fatti spiacevoli vi è sempre qualcuno che tira fuori la classica frase: «La violenza è figlia delle povere condizioni di vita della popolazione». Poi, in realtà, dopo qualche giorno, viene fuori dalle indagini che ad essere violenti non sono solo i poveri, ma anche - spesso e volentieri - i figli della buona borghesia. Per intenderci, a Catania e nel resto d'Italia esistono frange di violenti negli stadi: non tutti sono poveri e neppure tutti ricchi; la delinquenza esiste a prescindere dalle condizioni economiche. Negli anni si è lasciato crescere il fenomeno della tifoseria organizzata, una definizione quanto mai fuorviante, che fa da velo a gruppi di giovani ragazzi capeggiati spesso e volentieri da gente pregiudicata, che nulla ha a che fare con l'esercizio del tifo. Dopo ogni episodio di violenza, a prescindere dallo stadio e dalla tifoseria coinvolti, si sono sempre ripetute a vanvera frasi del tipo: «La stragrande maggioranza dei tifosi non è violenta»; «sono solo tre o quattro pseudotifosi»; «è poca gente a rovinare l'immagine di questa città» e altre banalità, mirate a difendere la squadra di propria appartenenza, la sua dirigenza e la zona geografica. Abbiamo sempre fatto in modo che a certi episodi non seguisse mai una severa e dura azione punitiva, affinché non vi fosse una prossima volta; l'istinto a coprire e a perdonare in nome di un generico tifo ha sempre avuto la meglio. Il perdurare di questo lassismo ha fatto sì che, al giorno d'oggi, interi settori dello stadio dello stadio siano in totale balìa di certe frange di tifosi violenti, che ormai fanno il bello e il cattivo tempo. È assolutamente insopportabile l'idea che per gestire 50 tifosi in trasferta occorrano 100 poliziotti sottratti all'abituale attività di *routine* per essere addestrati ad affrontare guerriglie urbane. Dal canto loro, gli ultras hanno propri gruppi fortemente strutturati, con confini ben precisi, in cui si condividono regole ferree e codici normativi ed esistono un *leader* carismatico, una simbologia condivisa (i colori della squadra), elementi di identificazione (cappelli, sciarpe, bandiere, eccetera). A tale percorso si è aggiunto, in questi ultimi anni, il progressivo radicamento di una violenza generalizzata, che trascende le rivalità prettamente sportive ed accomuna gli ultras in tutti gli stadi. Le tifoserie hanno oggi una base comune: non accettano più l'idea di alleanza, neppure su base politica; per questo motivo è nato lo *slogan*, sempre più in voga in tutti gli stadi, ma che

Solo questi dati sarebbero sufficienti a generare un forte allarme sociale, ma l'aspetto su cui i fatti di questi giorni devono farci riflettere è che la violenza a Catania, pur essendo ancora atipica, ha un obiettivo diverso da quello naturale: il nemico non era una tifoseria o una parte politicamente avversa, bensì era costituito dichiaratamente dalle forze dell'ordine e da tutto ciò che esse rappresentano, cioè le istituzioni e lo Stato. La dinamica diviene questa: noi tifosi, voi sbirri. Onestamente, non saprei quali possano essere state le contingenze che hanno portato a tale dislocazione dello scontro, ma sono convinto che sia necessario agire con la massima decisione per reprimere tali comportamenti pericolosissimi. Gli interventi legislativi per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi in questi anni sono stati numerosi, ma non sembrano aver risolto il problema, anzi, la violenza inizia a insediarsi anche nelle categorie minori; questo è dovuto, in parte, ad un cambio generazionale, ma anche al fatto che, spesso, le misure antiviolenza vengono aggirate. Non serve a nulla cominciare le partite con cinque minuti di ritardo, indossare magliette piene di *slogan*, utilizzare striscioni ed organizzare tavole rotonde. Per eliminare la violenza dagli stadi bisogna impedire che persone violente possano partecipare all'evento. Chi si rende protagonista di episodi di violenza deve essere allontanato per sempre dallo stadio. In estate, quando ancora il calcio è privo di valenza competitiva, gli stadi si riempiono di famiglie, non vi è separazione tra settori di tifosi e si vedono maglie di ogni tipo mescolate in tribuna, senza che accada nulla di pericoloso. Si pensi ai vari trofei triangolari marchiati da questa o quella bevanda: 60.000 persone insieme a condividere una festa senza correre alcun rischio. Questo dimostra inequivocabilmente che in assenza di gente violenta non c'è alcun timore di scontro tra tifosi di opposte squadre di calcio. L'odio e la stupidità non sono cose che si palesano allo stadio: chi è stupido e violento lo è sempre, chi non è violento non lo è mai, nemmeno in curva. Dinanzi ad episodi che costano vite umane non è più possibile tollerare i discorsi di coloro che tendono a difendere ogni manifestazione di libertà anche se si tratta della libertà di essere violenti. L'accento va posto sulle società calcistiche, che devono essere obbligate ad attuare tutti i necessari controlli per evitare che i giovani entrino negli stadi con oggetti pericolosi, oppure elaborare un piano efficace che agisca come deterrente ai comportamenti violenti e allontani le frange più intolleranti dei tifosi. Occorre senza dubbio rivedere gli stadi. Gli impianti italiani sono assolutamente inadeguati e le Amministrazioni comunali che ne sono spesso proprietarie non hanno le possibilità economiche di di intervenire per ammodernarli. Credo che sia giunto il momento di ripensare radicalmente il rapporto tra Comuni e società sportive. Le società devono prendersi l'onere di gestire anche la struttura in cui si svolge la loro attività. Per far questo, ovviamente, devono avere una ragionevole prospettiva

l'operazione economicamente sostenibile. In tale contesto vanno rivisti anche il ruolo e le funzioni che le forze dell'ordine devono essere chiamate a svolgere. Studi di sociologia hanno dimostrato che l'eccessiva visibilità delle forze dell'ordine in assetto antisommossa spesso finisce per ingigantire la proporzione della violenza. Ecco che allora l'acquisto degli impianti sportivi da parte delle società calcistiche e l'uso di personale interno, di strumenti di controllo a distanza sofisticati quali telecamere a circuito chiuso anche esternamente nelle immediate vicinanze degli impianti,

Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, con Catania si chiude forse definitivamente il sipario del lassismo, delle attese, di quel calcio romantico e popolare che ha attraversato questi anni difficili. La rivalità sportiva era diventata ormai un conflitto carico di veleno, una piattaforma gonfia di disprezzo, e di questo calcio malato si è detto molto, forse troppo, nell'ambito di queste ultime settimane. Sono stati accusati dirigenti e giornalisti, si è puntato il dito contro la nostra società che frustra i deboli e li spinge alla rivolta gratuita, si è riproposto l'oscuro intreccio tra tifosi e società, tra striscioni e scrivanie; ma tutto è stato inutile. Abbiamo probabilmente sbagliato le analisi, abbiamo probabilmente confuso lo spirito giustificazionista e assolutorio che il popolo del calcio innocentemente alimentava. In questo scenario gli stadi hanno perso progressivamente il loro pubblico e, soprattutto in questi ultimi anni, abbiamo assistito ad alcune sfide notturne che ci sono celebrate anche paradossalmente davanti a pochi intimi. Colpa delle televisioni, si è detto; bisogna prepararsi ad una società con poche migliaia di spettatori sugli spalti e con milioni di spettatori in poltrona. Eventi puramente mediatici, direi quasi da definire come satellitari. Ebbene, questo concetto si è oggi paradossalmente sublimato. Alcune partite si giocano infatti giustamente a porte chiuse e il tifoso è forzatamente ormai un protagonista da salotto, capace di vivere ogni sfida con la passione e il distacco di un rapporto lontano. In questo modo confuso, con la giostra dei tornelli, con gli stadi aperti agli abbonati, con provvedimenti certamente utili ma chiaramente parziali, il calcio ha provato a rimettere in piedi il suo tendone, provando soprattutto a riproporre la politica del *marketing* come unica icona contemporanea capace, spesso di coprire il teppismo, la violenza e in qualche caso anche la morte. Ma il pallone, nei nostri stadi, non può rotolare più con come una volta e questo decreto‑legge, nelle sue proiezioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza, fotografa una preoccupazione e determina svolte autentiche tutt'altro che formali. Lo ha illustrato puntualmente il senatore Sinisi in una relazione capace di individuare la tastiera degli interventi previsti. La riteniamo un'utile ed eccellente piattaforma di discussione, che merita certo ancora qualche limatura, ma che costituisce finalmente una risposta forte, vera, chiara e autentica ad una situazione non più accettabile e non più sostenibile. Una situazione che, probabilmente anche grazie all'applicazione più stringente del decreto Pisanu, può costituire una ricetta utile, una ricetta possibile per il calcio italiano. Un altro calcio è possibile,

del nostro sport. È un po' il riflesso, chiaro ed evidente, della nostra società: il denaro come unico riferimento certo e il prodotto capace di ammantare ogni problema, ogni incertezza. Ecco perché il fenomeno calcio andrà, da oggi in poi, costantemente monitorato: andrà monitorato nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Perché appare chiaro che il giocattolo ormai si è rotto e che la nostra società lo rende oggettivamente

le oscure connivenze, i falsi luoghi comuni che hanno caratterizzato il rapporto tra società e tifosi e l'elaborazione complessa del «sistema calcio». calcio». Credo che troppo spesso in questi anni la mancata applicazione di leggi esistenti, ma al tempo stesso anche un mancato inasprimento delle pene, abbiano finito per sviluppare una spirale assurda nella quale la parola «inedia» ha fatto troppo spesso rima con la parola «tragedia».

svolgere una riflessione chiara non soltanto all'interno di quest'Aula - come giustamente è stato fatto - ma anche attraverso una serie di audizioni che hanno coinvolto tutti gli attori istituzionali di questo processo. Riteniamo questo un primo importante momento per il Parlamento nel suo rapporto con lo sport italiano e ne avremo un altro nelle prossime settimane che sarà dedicato ai diritti televisivi del calcio, ad un altro fenomeno rilevante, che servirà probabilmente perché anche all'interno di quella realtà stiamo prevedendo interventi specifici connessi all'impiantistica sportiva. Segnerà probabilmente un altro fondamentale momento di riflessione e discussione per quanto riuscirà ad animare sul piano degli investimenti nell'ambito dell'impiantistica sportiva:

il rigore della discussione e la serenità con cui maggioranza e opposizione si sono confrontate rappresentano certamente un viatico ideale per costruire momenti di unione e al tempo stesso di riflessione comune rispetto a problemi che non hanno bisogno di bandiere.

desidero innanzitutto lodare la solerzia e la celerità con cui i due relatori Sinisi e Di Lello Finuoli hanno portato in Aula un tema di così scottante attualità. questo loro impegno, direi però che avevano ragione i nostri nonni: siamo in presenza del classico caso in cui chiudiamo la stalla quando i buoi sono ormai scappati, e sono scappati in due momenti. Il primo momento è sicuramente quello in cui

dell'emergenza dell'attualità nata dopo il caso di Catania. A questo proposito non bisogna mai sprecare occasione per rivolgere un pensiero deferente e affettuoso alla memoria dell'ispettore Raciti e soprattutto

i grandi proclami, le dichiarazioni commosse di personaggi di varia estrazione e diverso livello, anzi tutti di notevole livello, che sono sfumate di fronte a quella che per loro era la vera ed unica emergenza: emergenza: riaprire i botteghini degli stadi, riaprirli alle partite. Infatti, in poche settimane altro che blocco del campionato, sospensione di tre mesi e tutto quello che era stato proposto sullo slancio dell'emotività del momento! Tutto è ripreso come prima, ma fortunatamente per ora almeno non sul piano dei disordini. Sono stati quindi riaperti gli stadi; sono stati rilasciati molti degli indiziati dei gravi fatti di Catania; sono state ripristinate - è stato osservato - le partite serali; un generale rilassamento che è parente prossimo di una rassegnazione definitiva. Detto questo, in ogni caso non voglio vanificare lo sforzo dei relatori né l'importanza del disegno di legge in esame. Gli articoli 1 e 2 prevedono nuovi controlli, una prevenzione sicuramente più puntuale. Non dobbiamo però neanche nasconderci le difficoltà nel porre in essere queste previsioni, come per esempio quella sull'adeguamento degli impianti che alcune società hanno fatto in maniera rapidissima, miracolosa dopo anni e anni che se ne parlava. Abbiamo scoperto il miracoloso ruolo dei tornelli, di cui quasi tutti ignoravamo l'esistenza, che hanno risolto problemi

Quindi, non bastano controlli più severi e nemmeno l'inasprimento delle pene. La prevenzione va fatta mettendo con le spalle al muro e di fronte alle rispettive responsabilità i vari attori di questa scena: innanzitutto le società calcistiche, poi quelle che gestiscono gli impianti,

in stadi diventati improvvisamente bollenti per l'intolleranza e la sovranità garantita e tollerata delle tifoserie locali. In quel momento si trovava una soluzione tecnica per l'informazione ma si realizzava anche una grave sconfitta della legalità, che si arrendeva di fronte alla prepotenza. Mi auguro che questo decreto-legge risolva almeno il problema di restituire alla legalità anche il mondo del calcio, che è parte della nostra società e della nostra storia.

(«Le Temps») che mi ha fatto interrogare. Il titolo era «La tragedia del calcio mette in luce il lassismo delle autorità italiane».

perché «andare allo stadio con le tasche piene di bombe artigianali non è condannabile: il delitto sta nel lanciarle».

«oltre alla sua incommensurabile misericordia e al suo lassismo nei confronti dei delinquenti, il sistema italiano si caratterizza per il suo modo di propendere all'indignazione esagerata».

e della pericolosità del proiettile, che può essere un sasso che un tifoso scaglia contro un poliziotto fino ad ucciderlo

il lavoro svolto da parte delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, che hanno con intensità e rapidità lavorato ad un approdo unitario che considero particolarmente significativo. Da parte delle Da parte delle Commissioni e dell'Aula, tenendo conto degli interventi che ho ascoltato questa mattina, si è fino in fondo compreso

tesa a dare un segnale molto forte, un segnale di non sottovalutazione, di severità, che desse il segno che quella drammatica notte di violenza veniva immediatamente recepita come un punto di non ritorno, come un qualcosa cui dare risposte immediate, forti e inequivoche nel rispetto dei principi della legalità e della democrazia. Il decreto-legge oggi in sede di conversione è una misura urgente che tuttavia allude ad un disegno più di fondo: intervenire per rendere gli stadi più sicuri, per consentire che le manifestazioni sportive e calcistiche possano svolgersi in un clima di assoluta serenità, per permettere alle famiglie di ritornare tranquillamente negli stadi. esame allude a un disegno più di fondo, sul quale sicuramente il Parlamento sarà richiamato a discutere. Mi riferisco a quel disegno che dovrebbe portarci - questa è la mia opinione ad avere una netta distinzione tra la sicurezza interna agli stadi (che, da quel momento in poi, dovrebbe riguardare esclusivamente la società sportiva) e la sicurezza esterna agli stadi (che, invece, dovrebbe rimanere nelle disponibilità e nel lavoro delle Forze di polizia). È chiaro che tutto ciò allude al tema dell'impiantistica

una candidatura ufficiale del nostro Paese e che entro il prossimo mese di aprile sarà fornita al riguardo una risposta da parte degli organismi calcistici europei. Quindi servono un intervento urgente e misure più strutturali. Devo anche sottolineare che ci si è mossi

la decisa negazione di ogni deroga costituisca un punto fondamentale del decreto-legge.

che vede realizzare in tre giorni quello che precedentemente era previsto in sei mesi. Tutto ciò deve farci riflettere

La prima questione riguarda il tema delle trasferte dei tifosi, per le quali - ne avete discusso anche voi - spesso si impiega un numero spropositato di Forze di polizia. Il fatto che si stabilisca che le società ospitate abbiano il blocco dei biglietti da trasferire o da vendere ai propri tifosi costituisce un elemento fondamentale. In queste poche settimane di applicazione del decreto abbiamo registrato un abbattimento della presenza dei tifosi in trasferta del 90 per cento: se nelle settimane precedenti i tifosi in trasferta che si muovevano lungo il territorio nazionale erano 20.000,

radicalmente differente. Voglio soltanto segnalare un episodio che può apparire ai più particolarmente singolare, ma che invece è particolarmente rilevante per quanto riguarda le questioni dell'ordine pubblico. Ogni domenica, con le trasferte dei tifosi uno dei nodi fondamentali del controllo del territorio diventava il Comune di Villa San Giovanni, vicino Reggio Calabria. Ciò per una ragione semplicissima, cioè che lì passavano le tifoserie di quattro società di serie A: di serie A: la Reggina, il Palermo, il Catania e il Messina. Indipendentemente dal fatto che le squadre giocassero tra di loro, Villa San Giovanni costituiva un nodo da tenere in assoluto controllo, purché bisognava garantire che prima passasse la tifoseria del Palermo,

fossero Palermo-Messina, Messina-Reggina, Reggina-Catania o viceversa, e indipendentemente dal fatto che queste società poi giocassero a Siena, a Parma o in altre città del nostro Paese.

abbastanza incontrollabile di elementi di violenza. Nessuno può dimenticare, per esempio, che a queste trasferte spesso si accomunavano le devastazioni dei treni, degli autogrill, oltre ai rischi di incidenti negli stadi dove si svolgevano

Lo dico perché è stato sollevato il tema dell'articolo 6 e vorrei cercare di spiegare il testo del Governo; è chiaro che poi il Senato è sovrano e valuterà le mie argomentazioni. Noi affrontiamo nel decreto due questioni che considero fondamentali. La prima è l'interruzione di qualunque canale di collegamento economico tra le società sportive e le tifoserie. Sappiamo che questo è un elemento fondamentale,

che spesso ha portato ad un rapporto «non corretto» tra le società e le tifoserie, un rapporto in cui non era semplice identificare la vittima e il carnefice perché le parti si invertivano e ognuno pensava di poter controllare l'altro: le società pensavano di poter controllare le organizzazioni dei tifosi e queste di poter controllare le società. Con il decreto-legge viene vietato qualunque tipo di rapporto economico, anche nel campo del *merchandising*, e sappiamo quanto ciò sia importante. La seconda questione riguarda le misure di prevenzione personali e patrimoniali. Ho ascoltato qui le argomentazioni poste innanzitutto dal relatore e poi dai molti che sono intervenuti; voglio dire esplicitamente qual è il senso di questa norma. il senso di questa norma. Essa nasce da una questione che vorrei cercare di esplicitare sino in fondo e cioè che, nel momento in cui parliamo di violenza negli stadi, non parliamo esclusivamente dell'attività del singolo, ossia di colui che è artefice, attore di un'azione violenta. Noi vorremmo affrontare insieme con voi, in Parlamento, il tema delle organizzazioni dei tifosi. Non deve sfuggire a nessuno che questo tema è particolarmente complesso, perché sono organizzazioni cospicue, che risultano spesso avere rapporti con il mondo politico, con un mondo dell'estremismo politico, politico, ed hanno una struttura organizzata. L'articolo 6 consente di affrontare il tema del rapporto tra l'autore, l'attore materiale dell'atto di violenza, e coloro che organizzano queste strutture. Non sfugge a nessuno che dietro il fatto materiale ci sono coloro che hanno la possibilità di organizzare e - uso un termine forte - di utilizzare queste teste calde. L'articolo 6 consente di colpire, anche con misure di prevenzione personale e patrimoniale, coloro che utilizzano queste teste calde, perché sappiamo

Offre uno strumento di prevenzione in più; naturalmente è del tutto evidente che sto offrendo queste argomentazioni perché mi sono state esplicitamente richieste, ma il Senato è assolutamente sovrano. Non voglio convincere nessuno, ma non voglio neanche che passi l'idea che sia una norma assolutamente inutile. Dal nostro punto di vista essa ha una *ratio* (si può considerare quella *ratio* non sufficiente e tuttavia vorrei che fosse valutata per quello che effettivamente è): di comprendere l'evoluzione di alcune organizzazioni delle tifoserie, il rapporto che c'è tra coloro che compiono atti criminali e i favoreggiatori di quegli stessi atti, gli organizzatori, coloro che dirigono, che hanno in mano la struttura. Guardate, non c'è bisogno di particolari elementi di *intelligence*: se qualcuno di voi ha letto, per esempio, le interviste apparse in questi giorni sui giornali ai cosiddetti capi di alcune tifoserie avrà compreso che tipo di struttura e di organizzazione c'è dietro; basta leggere quelle interviste.

dal lavoro delle Commissioni, per due ragioni. La prima è che esso ci consegna un testo effettivamente migliorato nel merito;

e non sfugge a nessuno che il fatto che ci sia un sostegno unanime del Parlamento su questioni così delicate, che affrontano il tema del rapporto tra severità della norma e princìpi di libertà,

vorrei ritornare sulle considerazioni del vice ministro Minniti in relazione all'articolo 6 del decreto-legge, ossia le misure di prevenzione, perché nel corso del dibattito è sembrato che si volesse applicare alle associazioni sportive la legislazione antimafia. Sappiamo che non è esattamente così, nel senso che la legge n. 1423 del 1956, che si ritiene di applicare alle organizzazioni sportive, riguarda persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità; è la legge n. 575 del 1965 che ha ritenuto di dover applicare ai mafiosi la legge del 1956, non il contrario. Quindi le misure di prevenzione personale non riguardano i mafiosi: